la proroga di numerosi termini previsti da disposizioni legislative, con riferimento altresì a diversi ambiti settoriali (difesa, turismo, lavoro, salute, giustizia, trasporti, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e finanze). Si tratta di proroghe determinate dalla necessità di procedere ad un'adeguata e corretta attuazione di adempimenti di legge. Una seconda parte del provvedimento invece, disposizioni di carattere finanziario che intervengono in diversi settori: si tratta, in particolare, dei settori dei tributi, della borsa, dell'accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell'inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Altri articoli concernono altresì il trattamento del Fondo TFR e alcune norme relative alla violazione dell'obbligo delle comunicazioni nei confronti dell'ISTAT. La terza parte del provvedimento, infine, regola incentivi e contributi a favore di enti e soggetti diversi: si tratta di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare, alcuni finanziamenti. Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Vi sono poi norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

disposizioni in materia di adeguamento delle strutture turistico-ricettive alberghiere. Altre norme si riferiscono ai consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato e all'Unione accademica nazionale. Viene stabilita altresì una proroga per gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori licenziati della sanità privata e sono previsti termini per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte per i residenti del Molise e della Provincia di Foggia, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito quei territori. Vi sono disposizioni

corrisposto a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ. Ci sono anche norme che concernono le Regioni che non hanno perseguito tempestivamente nell'anno 2007 gli obiettivi programmati di risanamento e di riequilibrio economico e finanziario. Sono stanziati 250 milioni di euro per il Policlinico Umberto I e sono previste tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale. poi stabiliti termini per la predisposizione della rete nazionale delle banche dati per la conservazione dei cordoni ombelicali. Viene stabilito che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare è trasformato in Autorità nazionale per la sicurezza alimentare

sono norme che concernono il corretto funzionamento degli uffici giudiziari in mancanza di titolare, con la *prorogatio*per sei mesi dei titolari in carica.

La Presidenza del Consiglio viene abilitata a stabilire modalità di avvio di procedure per concorso pubblico e stabilizzazione di lavori flessibili. Questo termine viene prorogato al 30 giugno 2008. Vi sono poi una proroga dei termini per l'aggiornamento catastale

sulla pubblica amministrazione per l'accesso ai servizi in rete e limiti all'adesione dei Comuni a più forme associative comunali, norme in materia di autorizzazione integrata ambientale, di riscossione ed esenzione dal canone RAI per gli anziani,

concessioni di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili a responsabilità editoriale di emittenti televisive, norme sulle corse dei cavalli, riduzione del numero delle circoscrizioni per il decentramento comunale, l'attribuibilità del cinque per mille anche ad associazioni sportive e per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. Inoltre, sono previsti interventi per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, la sospensione dei termini tributari a favore di enti non commerciali che hanno una sede operativa in Molise, Sicilia e Puglia. una proroga per quanto riguarda i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia e norme concernenti le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza; e ancora, norme sulle istituzioni scolastiche che potranno riallocare le proprie risorse finanziarie. Viene previsto un termine per i rimborsi elettorali della legislatura che va a terminare. Viene stanziata anche una piccola somma per il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ci sono poi norme che concernono la Croce Rossa, che viene equiparata ad organizzazioni di volontariato. C'è una proroga al 31 dicembre 2008 per l'esenzione delle imposte di registro

l'università, la giustizia, le infrastrutture, i trasporti, il personale delle pubbliche amministrazioni, l'agricoltura, lo sviluppo economico, l'ambiente e gli affari interni. Il provvedimento, come si vede, è dunque diventato di natura estremamente complessa. È stato esaminato dalla 1a Commissione, affari costituzionali, molto rapidamente ieri mattina, con una buona intesa fra i Gruppi parlamentari, che hanno deciso di rimettere all'esame dell'Aula gli emendamenti presentati. presentati. In conclusione, voglio solo rassegnare all'Aula una evidente preoccupazione. Questo decreto-legge scade il 29 febbraio 2008. Oggi è il 27 febbraio 2008. La Camera credo debba essere convocata a domicilio. Noi siamo qui praticamente ad anticipare quella che potrà essere una riforma del Senato, che tutti quanti auspichiamo, e cioè che non ci sia un bicameralismo perfetto, perché

molte delle quali assolutamente rilevanti. Non posso dire che la Camera abbia fatto un buon lavoro, perché ci sono molte questioni che meriterebbero di essere risolte e altre che meriterebbero di essere espunte

a valutare con una certa comprensione l'esercizio rigoroso che dovrò svolgere nella funzione di relatore nel dare i miei pareri nei confronti degli emendamenti presentati. Quel che potrò fare è dare la mia

Signor Presidente, egregi colleghi, intervengo nel dibattito generale su questo provvedimento che è diventato, lo ha detto anche il relatore, l'ultimo treno per Yuma, un treno sul quale tutti disperatamente cercano di salire per salvarsi.

che, se fosse stata prevista in passato dai precedenti Governi, avrebbe innescato un'infinità di polemiche). È un provvedimento nel quale si ripristinano vecchie leggi; non solo si prorogano scadenze di leggi attualmente in vigore, ma si ripristinano vecchie leggi

(come se le caserme dismesse o da ristrutturare fossero solo a Bari, mentre sappiamo che ce ne sono decine e centinaia in tutto il Paese). Ma ho chiesto di intervenire soprattutto per una questione che riguarda la mia Regione. Il 13 e

che consente alla Regione di compartecipare al gettito dell'IRPEF derivante dai trattamenti pensionistici.

dello stanziamento di 30 milioni di euro anche per il 2010. Ma il problema di fondo è un altro. Nel Friuli-Venezia Giulia si contrabbanda questo provvedimento come un provvedimento che dal 2011 in poi consentirà alla Regione di godere di 200 milioni di euro l'anno ininterrottamente che potranno aumentare in base al gettito fiscale sulle persone fisiche derivante dalle pensioni. Ma ciò non è assolutamente vero. Mi dispiace che non sia presente il presidente della Commissione bilancio

Allora, capisco che l'ultimo treno per Yuma è un treno che dà anche tante illusioni, che deve creare tante illusioni al popolo, alla gente, consente di avere la speranza di salvarsi, di avere forse una prospettiva di ricchezza e di benessere. Però la gente non può essere imbrogliata, non le si può far credere che ciò che è in una legge corrisponde ad una cosa diversa rispetto a quella che viene venduta

una nuova norma e che questa non risolve assolutamente i patemi d'animo del presidente Illy. Quest'ultimo ha dichiarato sui giornali locali che, se il Senato non approverà la norma con questi soldi, egli non si candiderà. È da un mese mezzo che fa questo ricatto pubblico. Ma è possibile una cosa del genere? Non si sono mai verificate nella storia d'Italia situazioni di questo genere, in cui un governatore o un presidente locale ricatti il Parlamento nazionale per poter dare il via libera alla propria candidatura. La verità è che,

piccola questione che ho voluto sollevarle, è emblematico di uno strumento legislativo che forse andrebbe superato. Certo, siamo a fine legislatura e questo è l'ultimo treno che parte; quindi ognuno cerca di fare quello che può e di vendere il fumo che può. Però, onestamente, in questa nostra Italia non è più possibile continuare a creare illusioni oltre un certo livello all'opinione pubblica, perché immagino darà delle risposte assolutamente negative e di scarsa credibilità nei confronti della classe politica.

questo decreto-legge avrebbe dovuto rappresentare il corollario finale della manovra di bilancio, anticipata con il decreto fiscale. Una manovra di bilancio sbagliata nella sua impostazione di fondo, come dimostra l'andamento delle principali variabili economiche, sia quelle reali (minore crescita, maggiore inflazione, tanta smisurata pressione fiscale), che quelle di finanza pubblica, perché senza crescita non c'è risanamento. Oggi il Governo, ormai defunto, si presenta con questo atto conclusivo che dimostra il fallimento delle politiche finora realizzate, insieme al fallimento del Governo, al fallimento della coalizione, al fallimento dell'Unione e di tutto ciò che voleva unire l'impossibile. Si tratta di un decreto che non attiene solo a proporre in senso stretto, ma anche ad interventi legislativi che determinano un impatto sul quadro di finanza pubblica, con un peggioramento dei saldi e senza una reale valutazione degli effetti e dunque delle coperture.

La caduta del Governo ha impedito un ulteriore uso improprio delle risorse pubbliche. Mi riferisco al cosiddetto tesoretto, che potrà essere redistribuito solo dopo un accertamento serio delle maggiori entrate nel nuovo quadro quadro di finanza pubblica, così come determinato dalle variabili esogene. È evidente che un tale intervento non può essere adottato da un Governo inesistente, e questo lo dico perché ancora ieri il sottosegretario Grandi chiedeva un intervento in questo senso. Il Governo guidato da Prodi, nonostante due anni di crescita soddisfacente, ha condotto l'Italia al declino allontanandola colpevolmente dall'Europa.

Prodi, in sostanza, ha dilapidato due anni di crescita al 2 per cento e, soprattutto, un extragettito di 40 miliardi di euro, malamente sperperati sull'altare di controriforme delle pensioni e del lavoro. Basta ricordare quanto aveva ricevuto dal precedente Governo. A fronte di tale disastro, si approva, o si cerca di approvare, questo decreto-legge, che distribuisce prebende a destra e a manca, senza alcuna logica che non sia quella di tappare un po' di buchi laddove è necessario creare consenso clientelare, in vista della campagna elettorale imminente. Altro, presidente Morando, che «sportello Pomicino»: questo è ben altro! Basta leggere «Il Sole 24 ORE» di oggi, che parla di un peggioramento di 1 miliardo di euro. Per rendersi conto dell'impatto delle misure, basterebbe leggere le sempre attente analisi del Servizio bilancio del Senato,

pur se dimissionario, la dice lunga sugli imbarazzati silenzi ai quali stanno costringendo sempre più spesso la Ragioneria generale dello Stato. Per commentare solo alcune delle misure contenute in questo guazzabuglio di norme, si pensi al condono mascherato a favore dei concessionari e agli sconti ai Comuni protagonisti del disastro rifiuti in Campania. Invece di andare incontro al cittadino contribuente, vessato dalla cosiddetta multa pazza, si sceglie la strada opposta, ossia premiare i danni e gli errori prodotti dal sistema. Sono stati criticati i condoni del centro-destra: allora come si valuta la sanatoria della posizione dei concessionari, che hanno omesso di osservare l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento delle cartelle esattoriali relative ai ruoli consegnati prima del giugno 2008? Si tratta di una sanatoria retroattiva camuffata da deroga. L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle è un adempimento tassativo, previsto dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, lo statuto del contribuente,

le cronache abbiano stigmatizzato la scelta di sottrarre le società a controllo pubblico dal giudizio contabile della Corte dei conti, la norma è stata inserita in questo provvedimento. Ma era proprio necessario farlo in questo provvedimento o non era il caso di studiare attentamente il problema che certamente si pone sul doppio controllo, quello del codice civile e quello della Corte dei conti, per taluni tipi di società e per valutare attentamente quale dev'essere il limite da considerare? Allora, anche in questo senso, si è fatto scempio di una valutazione della Corte costituzionale. Ma il tempo è tiranno e mi limiterò ad altre, poche, considerazioni. Vediamo, per esempio, con soddisfazione che è stata affrontata la questione della rottamazione delle auto. La soddisfazione è doppia se penso ai veti opposti dai Verdi (ricordiamo quanto diceva il senatore Ripamonti in Aula ed in Commissione in opposizione a tale misura). Se guardiamo a ridurre concretamente le emissioni di CO2 nella prospettiva del 2012, rinnovando un vetusto parco-auto, è una misura necessaria. Non si fanno regali: si guarda ad adeguare l'impresa agli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Su nostra iniziativa è stata introdotta alla Camera una norma che consente la proroga vera dei termini per le dimissioni di quote di capitale eccedenti le soglie previste per le fondazioni bancarie al fine di favorirne il rientro e determinare le condizioni senza penalizzazioni. Non posso però, signor Presidente, non soffermarmi su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore: sulla vicenda dell'Ordine mauriziano. Un altro pasticcio si profila all'orizzonte: si passa da pasticcio a pasticcio. È il *de profundis* per l'Ordine mauriziano. Mi domando dove sono quelle forze che nella scorsa legislatura avevano posto questo problema ed, invece, oggi lo hanno dimenticato. Noi, al contrario, abbiamo assunto sempre posizioni limpide. limpide. Sapevamo che ci si sarebbe avviati verso un pasticcio legislativo fin dal decreto Pisanu, che abbiamo combattuto nella scorsa legislatura perché ha violentato una norma costituzionale. Credo che a questo punto la cosa migliore sia di cancellare la norma prevista dalla Costituzione. Vi sono responsabilità enormi da parte del commissario straordinario che ha gestito male l'intera vicenda, ma poiché le responsabilità sono anche politiche, esse non possono essere dissociate da chi ha determinato queste scelte. Allora, nonostante l'offerta di strumenti normativi efficaci, come abbiamo proposto nella scorsa legislatura, non si è levata alcuna voce. Il senatore Pisanu - mi dispiace che non sia presente - prenda atto della situazione e abbia il coraggio di fare autocritica e proponga di cancellare quella norma transitoria. In ambito fiscale abbiamo proposto, onorevole Lettieri, una proroga al 31 luglio 2008 per la consegna del modello 770 semplificato, in quanto vengono richiesti sempre maggiori adempimenti, sempre maggiori informazioni a carico dei soggetti come, per esempio, i codici fiscali dei familiari, le indicazioni dei dati per la verifica dell'erogazione del *bonus* degli incapienti e altro. Aumenta una burocrazia amministrativa che richiede un maggiore termine a disposizione.

Ma questa maggioranza si è piegata al veto di Rifondazione Comunista e, quindi, ha imposto sulla questione degli sfratti una soluzione anche dove non ve n'era bisogno. Altre questioni riguardano gli investimenti dell'INAIL, ma su questo ho presentato degli emendamenti. Non aggiungo altro, signor Presidente, se non la preoccupazione per un provvedimento che dilata ulteriormente la spesa e non determina le condizioni per il risanamento, nel silenzio di tanti rigoristi che in Aula si sono levati o si levano a giorni alterni e dovrebbero fare un pochino di autocritica nel momento in cui predispongono i programmi elettorali. finestra"). Assiste ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e di insegnanti del liceo ginnasio «Eugenio Montale» di Roma. Rivolgo a nome dell'Assemblea un saluto ai ragazzi e agli insegnanti. senatore Albonetti. Ne ha facoltà. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto 31 dicembre 2007, n. 248, il cosiddetto milleproroghe, è l'ultimo atto di una legislatura breve e combattuta, intensa e controversa; è il fotogramma finale che documenta un Paese che ha disperato bisogno di una trasformazione radicale, di interventi meditati e strutturali, ma che invece continua ad essere oggetto di semplici ritocchi, rinvii più o meno virtuosi, interventi di piccolo cabotaggio, il tutto con rigore *bipartisan*, l'unica forma di rigore cui sembra attenersi la politica italiana. Infatti, non c'è rigore finanziario in questo provvedimento, come ha dovuto riconoscere lo stesso Governo in Commissione bilancio quando sono stati discussi gli effetti sui saldi di finanza pubblica, e non c'è rigore politico, laddove non si porta a compimento quanto previsto dalla finanziaria all'articolo 1, comma 4, e cioè che tutto l'eventuale extragettito sia destinato a favore del lavoro dipendente.

che tra nuovi e vecchi partiti i fatti hanno preso il posto delle promesse. Non c'è poi un rigore etico, come si può constatare leggendo con attenzione i numerosi, troppi, articoli che riguardano interventi microsettoriali e/o microterritoriali. Del resto, il nomignolo "milleproroghe", da solo, allude ad una politica stagnante e incerta, fatta appunto di piccole cose, rinvii, accordi al ribasso, scambi su mercati minori. Ma, tant'è, criticata l'impostazione di fondo che nella prossima legislatura ci impegniamo a superare, possiamo indicare per titoli i provvedimenti che hanno un nostro consenso specifico in attesa di più coraggiose scelte strutturali.

le misure a favore di categorie deboli e che hanno contratto forti debiti di riconoscenza nei confronti dello Stato o aspettative di risarcimento (articoli 7-*bis*, 34-*bis*, 46 e 50). Infine, l'aumento di 16 milioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 13-*bis*) e gli interventi in materia di disagio abitativo (articolo 22-*ter*). sono i cardini attorno ai quali ruota il nostro consenso al disegno di legge. Sappiamo che molti cittadini italiani vogliono vedere e toccare ciò che la politica promette. Bene, l'articolo 22-*ter* riproduce quasi integralmente il disegno di legge dell'Atto Senato n. 1867 e sospende fino al 15 ottobre 2008 l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti di conduttori particolarmente disagiati, in attesa dell'attuazione del programma casa, conformemente alla legge n. 9 del 2007. La concreta difesa del diritto alla casa ha per la Sinistra Arcobaleno sufficiente cogenza per confermare, con un ultimo voto positivo, il vincolo sociale con tanti italiani.

il PD, il nuovo, Veltroni, che forse è da quarant'anni che calca le scene nazionali, se ne vergogni. Si vergogna di voi, probabilmente, di quello che avete fatto in questi due anni e non credo sia giusto. Lo dico perché agli avversari la Lega Nord riconosce la compattezza: in questi due anni avete fatto i salti mortali, siamo convinti che abbiate squassato il Paese, però, disciplinati, avete fatto il vostro dovere. Tuttavia,

Dobbiamo quindi ricordare ai padani e agli italiani questo disegno di legge con cui cercherete di fare la campagna elettorale. Il nuovo sostiene che non bisogna pensare al Governo, ma al Paese:

proroga ancora una bella trasformazione fondiaria di un bell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, il famoso EIPLI

Purtroppo, lascerete al prossimo Governo - e mi auguro per gli italiani e per i padani che non sia più il vostro - l'ennesimo buco e l'ennesima difficoltà.

apparentemente minimale in questo contesto così complesso e farraginoso che è il decreto milleproroghe: si tratta della proroga della nomina del Commissario straordinario del Governo per lo sviluppo del porto e della pertinente area di Gioia Tauro. È una nomina che non aveva ragion d'essere già in principio perché a Gioia Tauro c'è un presidente del porto e c'era il prefetto di Reggio Calabria, un brillantissimo funzionario che all'epoca hanno ritenuto non sufficientemente adeguato, salvo poi salvo poi cooptarlo nel Partito Democratico come capolista in Calabria (ma questa è un'altra storia). Ciò che veramente mi preme rassegnare all'Assemblea è la ragione sconcertante in forza della quale, con tre mesi di anticipo, si intende rinnovare una nomina che costa 600 milioni di euro l'anno e che dev'essere prorogata fino al 2009 a un personaggio assolutamente inutile, attesi gli assetti del porto di Gioia Tauro. Mi chiedo perché. È una vicenda come tante altre che si colgono leggendo questo documento

anche da alcune anomalie, signor Presidente, che è bene ricordare. Nel documento di sintesi che questo signore ha proposto all'Autorità portuale si è costituito un plagio. Questo signore percepisce tutti questi denari e beneficia di una serie di provvidenze e non è in grado di redigere un documento organico nel quale possa trasfondere il proprio pensiero e dare degli impulsi

di grottesco papello che non servirà a nulla ma è utile soltanto a questo signore, ai suoi amici e agli amici degli amici. Ebbene, un simile personaggio vuole essere prorogato. Mi auguro che l'Assemblea abbia un rigurgito di dignità e questo punto lo bocci clamorosamente.

che il provvedimento milleproroghe su un tema molto importante per il futuro del nostro Paese e cioè l'università e la ricerca sia la testimonianza del fallimento della politica universitaria di questo Governo.

è tornata perché questo Governo, in due anni, non solo non ha saputo applicare la legge Moratti, nonostante l'opposizione si fosse dichiarata disponibile, eventualmente, a prendere in considerazione

di siffatto provvedimento e puntualmente, la Corte dei conti, recependo tutte le indicazioni che noi avevamo denunciato, lo ha dichiarato assolutamente illegittimo. In questo contesto devo dire che amareggia vedere come norme di dieci anni fa, che erano state superate nella passata legislatura con il ritorno ad una più seria forma di reclutamento nazionale,

consentiva di destinare il 30 per cento delle risorse a quelle università che avessero raggiunto risultati significativi in tema di ricerca e di didattica. Quell'emendamento venne bocciato. Inoltre voglio aggiungere che questa maggioranza e questo Governo

è una componente dell'attuale Partito democratico al Governo che ha una responsabilità fondamentale per aver voluto a tutti i costi un Regolamento, quello sui ricercatori, che ha impantanato la politica governativa sull'università, impedendo una riflessione seria, serena, anche nel dialogo con l'opposizione per una riforma forte del sistema universitario. Ho apprezzato l'ordine del giorno che il relatore Ranieri ha presentato ieri in Commissione e che abbiamo approvato all'unanimità.

sollevare una questione in materia di gestione dei rifiuti, problema affrontato da questo decreto. Accogliendo l'invito del relatore Sinisi a non formulare emendamenti, dati i tempi a disposizione,

«Il comma 3 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente: "non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se trattati, in fognatura"». Fin qui va tutto

(«Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura»). A conferma che trattasi di errore di mancato coordinamento, nella nota 2 all'articolo 2, pubblicata a pagina 55 della stessa *Gazzetta Ufficiale*

risulta il seguente testo del comma 3: «Non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura». Quindi, correttamente, il mantenimento del testo del citato comma 19 dell'articolo 2. Tale erroneo mancato coordinamento sta ingenerando dubbi interpretativi con conseguenze rilevanti, non tanto sui rifiuti triturati in fognatura, ma su altri rifiuti (per esempio quelli liquidi) che, anche se pretrattati e specificatamente autorizzati, non potrebbero a mio parere, non dovrebbero - essere sversati in fognatura. Chiedo al Governo la cortese attenzione intanto per confermare in questa Aula tale interpretazione, che io ritengo corretta ed evidente,

assomiglia molto al cestino della carta straccia che alla fine della legislatura, anziché essere buttato, è stato ripescato e rischia di diventare legge. Tale eventualità, a mio avviso, sarebbe alquanto pericolosa, anche perché sotto il profilo finanziario, questione

non è pensabile che la copertura si rifaccia all'andamento della situazione macroeconomica, dato che essa non è brillante come in precedenza, che l'economia ristagna, l'euro si apprezza di valore e che il petrolio cresce di prezzo. Quindi, i dati del 2008 non sono allo stato attuale particolarmente confortevoli. Una serie di misure contenute nel decreto, inoltre, aggraveranno sicuramente la spesa, perché molte coperture sono state

si tratta di spese sostanzialmente non coperte. Vi è poi tutta la vicenda dei concessionari e l'abolizione dell'obbligo di versamento di 4,6 miliardi per il 2008, coperto con l'obbligatorietà del trasferimento del TFR da parte dell'INPS per una cifra equivalente nel 2007; ciò si traduce in un buco nel 2007 per quanto riguarda l'indebitamento, buco che in ogni caso

il senatore Valditara ha parlato a lungo dei limiti dell'azione del Governo in materia di ricerca e università.

una delle ragioni fondamentali delle politiche di scambio nella selezione dei docenti universitari effettuata dalle università italiane. italiane. Tutti i rettori delle più importanti università italiane hanno affermato che tale meccanismo mette in discussione la capacità delle università di programmare i propri organici e i propri conti economici.

aspetto. Tutti parlano di bipolarismo mite e personalmente sono da sempre un sostenitore di un bipolarismo che non eviti il confronto di merito,

oppure un bipolarismo mite, che affronta il merito dei problemi e fa accordi unicamente in funzione del rinnovamento, dell'innovazione e del miglioramento del nostro sistema universitario e di ricerca. Nella

Presidente, in sede di replica intendo soltanto accogliere la precisazione fatta dal senatore Ronchi. In effetti si è creato un disordine normativo nel momento in cui una norma abrogativa è stata ritenuta, inopportunamente e incautamente, in vita nel testo che era stato presentato. Tuttavia la nota di ripubblicazione della legge in questione, riguardante la possibilità di ammissione in fognatura di taluni rifiuti triturati,

discussione di questo decreto-legge non consente di intervenire qui con una precisazione in tal senso, ma credo che l'interpretazione della volontà del legislatore ed anche la chiarezza della norma dovrebbero

agli onorevoli senatori che è prassi necessitata l'emanazione di un decreto di fine anno. Per dare continuità all'amministrazione i Governi *pro tempore* (non solo questo, ma anche quelli che lo hanno preceduto) da tempo adottano lo strumento della decretazione di fine anno. Il testo originale

ha accolto molti emendamenti sui quali, oggettivamente, sussistevano elementi di criticità e di perplessità. Ora non c'è più tempo per consentire al Senato di espungere e modificare le norme che non sono del tutto organiche. Comprendo, quindi, le critiche che sono venute e faccio appello non al bipolarismo mite, ma al bipolarismo intelligente, al senso di responsabilità, alla comprensione

ai provvedimenti relativi alla rottamazione, che possono contribuire al rilancio della nostra attività imprenditoriale. Penso alle norme relative ai rifiuti, con il dramma che sta vivendo la Regione Campania, agli interventi previsti per gli ammortizzatori sociali nell'area di Malpensa, con il problema dell'assegnazione degli *slot* legata alla vicenda Alitalia e ai finanziamenti previsti per le opere pubbliche in quell'area. Certo, nel provvedimento vi sono norme che

Penso ancora a norme che andavano inserite per consentire, per esempio, l'accatastamento degli immobili rurali, come chiesto da moltissimi Comuni, o a provvedimenti aventi un forte impatto sociale, quale la proroga degli sfratti, che è stata necessitata a seguito di un disagio abitativo in molte aree, soprattutto metropolitane. Vi sono interventi finalizzati, ripeto, allo sviluppo. Ho parlato della «Visco Sud», ma vi sono anche quelli relativi agli investimenti degli enti previdenziali per costruire, per esempio, la cittadella della polizia in Campania.

Sento il dovere di fare appello al Senato perché consenta l'approvazione definitiva di questo provvedimento. Il dibattito, cui ho prestato doverosamente attenzione, è stato ricco e alcune critiche sono - ripeto - comprensibili ma ricordo che alla Camera - questa è la verità, senatore Vegas - il Governo non ha presentato alcun emendamento. Tutte le modifiche sono di origine parlamentare

suprema del Senato, questo deve essere chiaro, ma l'aspetto politico non può essere sottovalutato né ignorato. Circa il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, mi corre l'obbligo di ribadire in questa sede che il provvedimento, in termini di saldo netto, non costa, o meglio, esso va tutto sulla riduzione di autorizzazione di spesa o sul ricorso al fondo speciale, cioè alle Tabelle A e B della legge finanziaria. Anzi, c'è un lieve saldo attivo: 43,8 milioni per il 2008; 67,9 per il 2009; 161,9 per il 2010. Qualche problema potrebbe esserci per l'indebitamento relativo al solo 2008, ma anche su questo punto devo precisare che, per qualche spesa, nel caso dei 500 milioni previsti a carico degli enti previdenziali, la stima è stata prudenziale,

Relativamente ai 4,6 miliardi di euro del mancato acconto dovuto dai concessionari della riscossione e, in particolare, alle preoccupazioni per la sua mancata copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, faccio notare che tale cifra è riassorbita nel miglior andamento dei saldi di finanza pubblica. È vero che il provvedimento non poggia, così come è stato evidenziato correttamente nella Commissione bilancio, bilancio, la propria valutazione su una revisione formale delle previsioni di finanza pubblica, ma occorre tener conto che il Ministero dell'economia e delle finanze svolge una continua e costante azione di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, che consente di verificare in qualsiasi momento il reale andamento dei conti. Sottolineo poi che la cifra di 4,6 miliardi è pari a circa lo 0,3 del PIL. è pari a circa lo 0,3 del PIL. Vi è quindi la possibilità di chiudere il consuntivo 2007 con un livello di indebitamento migliore di quello a suo tempo programmato (2,4 per cento), attestandosi complessivamente intorno al 2-2,1 per cento. Quindi, nonostante l'effetto negativo della disposizione di cui sta discutendo, il conseguimento dell'obiettivo, in termini di indebitamento netto, ci sarà. In questo senso il maggiore fabbisogno di cassa può ritenersi compensato. Naturalmente, questo allo stato degli atti. Per il futuro gli scenari sull'andamento dell'economia mondiale, dell'Eurozona e - se volete - del nostro Paese in particolare non sono confortanti; basti considerare l'aumento quotidiano del prezzo del petrolio, del grano, il rapporto dell'euro con il dollaro e con altre monete. Sono tutti elementi che suscitano preoccupazione. Ciò nonostante, dobbiamo avere fiducia nella capacità del sistema Paese, del nostro mondo imprenditoriale e, mi sia consentito, anche anche nella bontà delle decisioni che spetteranno al nuovo Parlamento e al nuovo Governo. Nel ringraziarvi rinnovo l'appello a ritirare tutti gli emendamenti; eventualmente quelli verso i quali

che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti che non riguardano proroga di termini o che tendono ad introdurre materie nuove rispetto al testo del decreto-legge come trasmesso dalla Camera dei deputati. Sono altresì inammissibili proposte emendative che modificano in modo frammentario o parziale atti di rango normativo non primario. Ricordo che il vaglio di ammissibilità della Presidenza riguardo agli emendamenti presentati sarà particolarmente rigoroso, tenuto conto dello svolgimento dei lavori parlamentari in regime di *prorogatio* e della particolare posizione costituzionale di fronte alle Camere di un Governo dimissionario. Risultano pertanto inammissibili i seguenti emendamenti: 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6-*bis*.100 (seconda parte), 6-*quater*.0.101, 7-*bis.*0.100,

La Commissione osserva inoltre l'opportunità che nella valutazione della copertura delle singole leggi di spesa sia assicurata la compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., in quanto in quanto si può ritenere che l'attuale sistema di regole (anche conformemente a quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006) non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione di tali effetti. In relazione all'articolo 29, recante incentivi alla rottamazione, la Commissione osserva che la metodologia di stima degli effetti indotti positivi si pone in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi in occasione della quantificazione degli effetti di analoghi provvedimenti di agevolazione. L'utilizzo a fini di copertura delle maggiori entrate derivanti da norme agevolative (cd. effetti indotti) dovrebbe, peraltro, essere limitata alla sede della manovra annuale di finanza pubblica, nella quale le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica sottostanti al quadro programmatico inglobano gli effetti complessivi associati all'azione del Governo, laddove in sede di stima delle singole misure sussiste il rischio di non tener conto di tutti i complessi canali di retroazione che interessano il sistema economico, determinando la duplicazione di effetti finanziari positivi ovvero trascurando effetti di sostituzione di segno opposto. In relazione all'articolo 36, recante soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, la Commissione osserva che la mancata copertura degli effetti finanziari per l'anno 2007 (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) in quanto ritenuti riassorbiti nell'andamento di finanza pubblica più favorevole rispetto alle previsioni iniziali e quindi coerente con gli obiettivi programmatici di cui al Patto di stabilità e crescita, essendo avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non sembra in grado di fornire una garanzia della tutela degli obiettivi programmatici di finanza pubblica». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 36-*bis*.0.100, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.101, 3.102, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105,

Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 24-*sexies*.0.101 nel presupposto che i contratti di lavori flessibili vengano stipulati nell'ambito delle risorse assegnate e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Presidente, ho ascoltato gli *speech* che sono stati letti dalla Presidenza, per quanto riguarda le inammissibilità, e dal segretario addetto alla Presidenza, il collega senatore Malan, per quanto riguarda i pareri della Commissione bilancio. Presidente, mi consenta di svolgere due considerazioni. In primo luogo, per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, laddove si stabilisce quali siano gli emendamenti per i quali viene espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarebbe preferibile che venisse specificato, così come fa la Presidenza, anche il titolare o il primo presentatore dell'emendamento, in modo che si riesca, pur nel vortice di una seduta che deve essere rapida e probabilmente non esaustiva (se non per alcuni), a comprendere quello di cui stiamo parlando. Sulle questioni sollevate, signor Presidente, voglio che resti a verbale che prendo atto di come ci sia stata, oltre alla modifica della legge elettorale (e sappiamo tutti come), anche la modifica di quello che era uno dei cardini del nostro ordinamento: il sistema bicamerale perfetto. Perché? signor Presidente, nel momento in cui si consente alla Camera di stravolgere un decreto-legge nel quale è stato infilato di tutto, un decreto‑legge che da "milleproroghe" diventa "millemarchette", senza confini e senza decenza alcuna,

È molto più. Allora, scusatemi, c'è una prerogativa che va tutelata o difesa. O qualcuno ha il coraggio di dire che è preferibile che nessuno parli e che quindi gli emendamenti presentati decadano (un poco perché vengono dichiarati inammissibili dalla Presidenza, un poco perché c'è la contrarietà della Commissione bilancio), oppure non ci si venga a dire che, in queste condizioni, i limiti entro i quali vanno presentati gli emendamenti sono quelli che riguardano soltanto la proroga di termini o che introducono materie nuove. Presidente, mi affido alla sua saggezza, non ho bisogno di insistere su questo punto. Questo decreto-legge

Presidente, la questione è ancora più grave, per una motivazione molto semplice. Nel momento in cui era in discussione un altro decreto-legge molto delicato, quello sull'*election day*, che in qualche modo toccava i diritti e le prerogative pretese e presunte dei partiti, qualcuno, da un Colle molto alto, ha preteso di intervenire perché si ristabilisse una correttezza e un rispetto costituzionale. In quel caso erano lesi gli interessi e i diritti dei partiti, ammesso che fossero lesi (su questo ho un concetto molto diverso: o la deroga valeva per tutti o non aveva diritto di cittadinanza e non doveva valere per nessuno). Detto questo, c'è stato un intervento al quale tutti ci siamo inchinati e adesso che invece è in discussione un decreto millemarchette, che tocca la finanza pubblica, la spesa e la gente, quali interventi registriamo? Chi controfirmerà un provvedimento del genere, dove solo per decenza la Commissione bilancio dichiara la sua contrarietà? Sapete che cosa contiene il provvedimento in esame? Io illustrerò tutti i miei emendamenti e chiederò che vengano sottoposti al voto elettronico, perché spero che ci sia la consapevolezza di quanti preferiscono sfuggire o sottrarsi alle responsabilità, a cominciare dal relatore. Tuttavia, Presidente, c'è un problema complessivo di agibilità democratica. Non possiamo pretendere che ci sia il rispetto delle norme e degli interessi, che hanno comunque un'interfaccia nella Costituzione in alcuni momenti, e poi essere quantomeno sciatti, se non corresponsabili di atteggiamenti come questi, che veramente ci mettono in condizione di doverci vergognare di quello che stiamo facendo. facendo. Illustrerò gli emendamenti nel merito; invito i colleghi a leggere solo i titoli delle norme che sono state introdotte alla Camera e a valutare se sia comprensibile ed accettabile che dallo scranno più alto del Senato ci venga la seguente indicazione: non potete che presentare alcuni emendamenti. Usciamo allora dalla farsa, anche perché siamo alla fine di una recita che probabilmente non ha soddisfatto nessuno, né quelli che vivono qui dentro, né quelli che vivono fuori. Cerchiamo di essere una volta tanto

da quelli del Senato, perché si tratta di modifiche che sono state sostanzialmente accettate da tutti. Aggiungo che stiamo trattando questo provvedimento a Camere sciolte e con il Governo in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione. È di solare evidenza che, laddove vi fossero delle modifiche, la conseguenza non sarebbe l'approvazione della modifica, ma la decadenza dell'intero provvedimento, mentre ci sono molte misure che meritano di essere accolte. Voglio ricordare soltanto la questione dei rifiuti solidi urbani a Napoli e la tragica emergenza che va affrontata insieme a tante altre iniziative che servono a questo Paese affinché possa affrontare i disagi che certamente ci saranno per la mancanza delle istituzioni nella loro piena funzionalità nei prossimi due mesi fino alla

L'argomento in questione è oggetto di dibattito, di valutazione ed è all'ordine del giorno il problema della detassazione dei salari e degli stipendi. Vi è un problema di giustizia sociale che il Governo Prodi aveva già affrontato, avviando incontri con le forze sociali ed impegnandosi con trimestrale di cassa, a valutare le reali disponibilità per procedere in quella direzione. Perciò esprimo parere favorevole all'ordine del giorno che ritengo si faccia carico di sollevare una questione di enorme attualità. Come ha fatto il relatore, esprimo anch'io parere favorevole su tutti gli altri ordini del giorno, così come modificati su indicazione della Presidenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero di grande rilievo che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno G100. Mi auguro, però, che alle parole seguano i fatti. Nel dibattito alla Camera dei deputati il Partito Democratico ha aperto una polemica con il Popolo della Libertà perché il Partito Democratico ritiene che un provvedimento, come quello da noi chiesto - almeno così ha fatto alla Camera - possa essere approvato solo con l'intesa dell'opposizione, prefigurando così quello che già si intravede all'orizzonte, dopo le prossime elezioni.

sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti

Quindi confidiamo sulla serietà di questo impegno, con cui si chiede al Governo Prodi di emanare tale anche in questa fase, dinanzi ad una vera e propria emergenza sociale, come quella della perdita del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, dei ceti popolari e della povera gente, che l'ISTAT ha quantificato giustamente indicando l'indice del costo della vita per i prodotti che abitualmente i cittadini consumano tutti i giorni.

I sindacati e le forze sociali chiedono con grande determinazione che a questo si provveda. Se la dichiarazione è seria, come non ho ragione di dubitare, chiediamo che, al prossimo Consiglio dei ministri, il Governo emani un decreto-legge con il quale predisporre una prima detrazione, come chiede il nostro ordine del giorno, per i redditi da lavoro dipendente più bassi, salvo stabilire con provvedimenti successivi, e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo stanziamento definitivo per tale detrazione. È una proposta seria che rientra perfettamente nei binari istituzionali e nelle compatibilità di bilancio. Nel momento in cui tutti promettono mari e monti a destra ed a manca, ci aspettiamo dal nostro Governo, come suo ultimo atto, una misura indispensabile di risarcimento sociale.

con una ristrutturazione nel settore automobilistico che inizia con qualche anno di ritardo. Ma quei lavoratori operai della Ford guadagnano 80.000 dollari l'anno; un lavoratore operaio nel nostro Paese guadagna 20.000 euro l'anno. Questa è la condizione del lavoro salariato nel nostro Paese. Paese. Ho chiesto di intervenire perché non resti sotto silenzio il fatto che la Presidenza abbia deciso di non considerare ammissibile un ordine del giorno che chiedeva che fosse rispettata la legge finanziaria. È inammissibile che il Senato non possa discutere del lavoro e della sua condizione. È inammissibile che il Senato non possa discutere del valore del lavoro in questo Paese, con le condizioni

Credo che nel tempo che resta al Senato le Commissioni debbano lavorare per dare certezza affinché quella legge, che segna un punto di avanzamento e di civiltà sulla questione della sicurezza del lavoro, diventi operativa.

una loro capacità di rappresentare un momento di sofferenza autentica, sono negli ordini del giorno. Siamo arrivati purtroppo a questo punto. L'ordine del giorno affronta un'emergenza reale pretende un intervento cogente, immediato, come, d'altra parte, già previsto nella finanziaria. Certo, riteniamo che l'intervento in questa materia sia, di solito, abbastanza complicato. Sia se si utilizza la leva fiscale, sia se si utilizza la leva retributiva per cercare di operare un recupero del potere di acquisto dei salari, in ogni caso il problema che quando non si interviene sul controllo delle dinamiche dei prezzi, alla fine, tutto può rimanere abbastanza inefficace.

sulla questione dei rifiuti. Mi rendo conto che i rifiuti in Campania sono serviti a fare in modo che qualcuno accumulasse tanta ricchezza; sono riusciti a nascondere tanti disagi. Anche il Governo e il relatore utilizzano i rifiuti per nascondere tante marchette che sotto quei rifiuti sono depositate. Mi sembra un atteggiamento molto discutibile di chi, invece, avrebbe potuto coltivare per per strade separate la possibilità di approvare provvedimenti che non operassero un effetto di trascinamento rispetto a norme che nessuno in questo consesso conosce, ma che domani riverbereranno effetti negativi sulla nostra società.

direttamente dalle previsioni dell'ordinamento giudiziario. Quindi significa allineare con la normativa vigente una previsione che diversamente risulterebbe completamente sfasata.

per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003. Eppure, signor Presidente, sia il servizio studi della Camera sia chiunque si apprestasse a leggere il provvedimento verificherebbe che non appare assolutamente chiara la portata normativa di tale ultimo riferimento proprio perché ai commi 19 e 22, della legge finanziaria non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate. Cioè si opera un differimento per consentire una devoluzione che in effetti non è prevista chiaramente.

in questo decreto una modifica sostanziale della responsabilità contabile degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, provocando un effetto contrario a quello che noi oggi dobbiamo perseguire, ossia quello di un rafforzamento delle forme di responsabilità. Dobbiamo infatti tutelare meglio la corretta gestione del denaro pubblico. Questa è una norma adottata palesemente sulla spinta di *lobby* potenti, così come anche l'altra sulla proroga della durata delle Autorità. Non sono queste le cose che si possono fare decentemente nottetempo in un provvedimento normativo di questo genere. Ripeto, ritiro l'emendamento per non

l'introduzione dell'articolo 16-*bis* sostanzialmente si esclude la responsabilità erariale, quindi la verifica ed il controllo della Corte dei conti, per alcune società a partecipazione pubblica. È una di quelle marchette nascoste in questo decreto, perché in qualche modo si rendono irresponsabili alcuni amministratori di società con prevalente interesse pubblico. È assurdo che una norma come questa passi sotto silenzio.

Voglio sapere quanti e quali colleghi sono per concedere un regime di irresponsabilità a società a prevalente controllo pubblico quotate in borsa. Questo il senso dell'emendamento che mantengo e per il quale chiedo la votazione con sistema

più accettabile il clima in magistratura poiché è evidente che coloro i quali hanno già compiuto gli otto anni e devono lasciare gli apici della magistratura o accettano di andare chissà dove e chissà come, oppure sono costretti a rimanere in soprannumero nell'ufficio nel quale attualmente risiedono ed è evidentemente assurdo che colui il quale ha rivestito l'incarico di procuratore capo, per esempio, accetti di rimanere nella stessa procura in una posizione di soprannumero e chiaramente

che si esprimono quotidianamente su problematiche che riguardano la giustizia valutassero concretamente la portata di questo emendamento che cerca, signor Presidente, di sventare le conseguenze già anticipate da alcune decisioni (mi riferisco, per esempio, al TAR del Piemonte che ha lasciato intendere come proprio perché ci sono stati già dei ricorsi occorre mettere in campo delle contromisure). Questa è, appunto, una contromisura che restituisce dignità ai magistrati ed evita ulteriori conseguenze. Se qualcuno la vuole condividere o commentare ne sarei lieto visto che i limiti temporali a mia disposizione, purtroppo, non me lo consentono. Su

qui presente il Ministro della giustizia. Ebbene, signor Ministro, se lei all'esito del mio intervento formulerà un invito al ritiro dicendo evidentemente che quello che affermo non corrisponde al vero, io ritirerò l'emendamento.

il secondo comma dell'articolo 16‑*ter*, il quale, con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari di Bolzano, cancella una norma dell'ordinamento giudiziario

gli uffici giudiziari d'Italia. Il che equivale a dire che nella Provincia di Bolzano i giudici possono passare da pubblico ministero a giudice e da giudice a pubblico ministero nello stesso identico ufficio giudiziario. Primo punto, signor Ministro: a me pare che questa sia una intollerabile disparità di trattamento. Davvero non comprendo la ragione per la quale tutti i giudici d'Italia devono passare distretto se vogliono cambiare le funzioni, mentre invece solo ed esclusivamente i giudici degli uffici giudiziari di Bolzano possono passare dall'ufficio del pubblico ministero all'ufficio del giudice nello stesso identico circondario, senza neanche recarsi nel circondario di Trento, limitrofo, com'era previsto nell'ordinamento giudiziario. Seconda cosa che mi permetto di dire, con l'abrogazione di questa norma la questione dei passaggi di funzione da requirente a giudicante è completamente sprovvista di disciplina. vero, infatti, che nel secondo comma dell'articolo 16-*ter* si fa riferimento all'articolo 2 della legge 150 del 2005, ma ella sa, signor Ministro, che quella norma è la legge delega dell'ordinamento giudiziario, una legge che è stata compiutamente esercitata, che si è caducata con l'esercizio delle deleghe e che, in ogni caso, non ha alcuna natura precettiva. Allora, signor Ministro, in conclusione, le chiedo di volermi smentire su questo e, se lei lo farà, io ritiro l'emendamento: è vero o non è vero che, a seguito di questa norma, i magistrati degli uffici giudiziari di Bolzano avranno un trattamento completamente diverso dai magistrati di tutti gli uffici giudiziari d'Italia? È vero o non è vero che la norma che rimane, cioè quella della legge delega, non ha natura precettiva e che conseguentemente, in ragione dell'assenza della natura precettiva di quella norma, non vi è una disciplina che regolamenta il passaggio di funzioni da requirente a giudicante e da giudicante a requirente solo ed esclusivamente per i magistrati degli uffici giudiziari di Bolzano? Aspetto la sua parola per decidere.

vorrei segnalare la delicatezza della questione di cui stiamo parlando. Se il Governo, dopo l'accoglimento degli ordini del giorno da noi presentati, non interverrà stanziando le risorse adeguate

per mantenere in esercizio l'attuale livello di servizio per le Regioni. Il Governo, all'epoca, non identificò le risorse, ma si impegnò a trovarle successivamente.

Purtroppo questo provvedimento, pur ampliato a dismisura, non contiene tali risorse. Pertanto, chiedo e prego il Governo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime ore di trovare la soluzione, altrimenti ci sarà giustamente - io naturalmente sarò al loro fianco avendo combattuto pienamente - la rivolta dei pendolari, che chiedono servizi migliori e di qualità e, come risposta, si vedranno chiudere gli attuali livelli di servizio. Si tratta quindi di una questione delicatissima sulla quale chiedo da parte del mio Governo (per quanto esso abbia concluso la propria esperienza) la massima attenzione, per garantire ai cittadini e alle cittadine italiane un servizio di qualità mantenendo almeno l'attuale livello di treni pendolari. intervengo solo per una precisazione che fa riferimento all'ordine del giorno G21-*quater*.100, ma vale per tutti gli ordini del giorno. Come ha detto il presidente Marini all'inizio della seduta, gli ordini del giorno sono degli inviti al Governo, perché il Governo è in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione. Siccome in alcuni testi si afferma "il Governo garantisce" e "il Governo si impegna", è chiaro che tutte queste evocazioni valgono come invito ed esortazione al Governo. PRESIDENTE. Gli uffici li hanno predisposti sotto questa forma.

Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino) nei quali la legge n. 9 del 2007 ha prodotto più di trenta sfratti bloccati. È lì che esiste un problema abitativo che occorrerebbe risolvere. La vittoria di Rifondazione Comunista all'interno della coalizione ha imposto un blocco generalizzato anche dove questa emergenza abitativa non c'è. Nella predisposizione di programmi che si sta operando, sia da parte di partiti del centro‑destra che del centro‑sinistra, viene posto il problema del mercato, della libera contrattazione, del rilancio delle politiche abitative, delle cedolari secche, delle imposte sostitutive: dopo però procediamo in questo senso, che è illogico e contro il buonsenso. Siamo favorevoli ad intervenire laddove c'è necessità e non dove non c'è alcuna necessità. Per queste ragioni, signor Presidente, invito l'Assemblea a votare questo emendamento e chiedo il supporto della votazione elettronica.

i piani secondo quanto viene indicato, cioè con tassi di rendimento del 3,1 per cento del capitale investito. Allora, propongo e sollecito l'attenzione affinché siano portate a compimento le istruttorie, quanto meno quelle già avviate di particolare rilevanza sul piano sociale. È una mera indicazione per richiamare la contraddizione di questa norma soprattutto con riferimento ai fondi immobiliari che hanno necessità di intervenire e di realizzare introiti coerenti con l'investimento in termini di mercato.

Naturalmente vogliamo ribadire anche in questa sede di dichiarazione di voto la nostra contrarietà più assoluta, invitando l'Assemblea ad una riflessione: è veramente sperpero di denaro pubblico quello che si sta realizzando in questo momento. Auspico pertanto un recupero di dignità da parte dell'Assemblea perché si possa evitare questo sconcio.

Signor Presidente, come i colleghi avranno verificato, poco fa mi sono rivolto all'Assemblea chiedendo che qualcuno mi desse la possibilità di continuare a parlare, visto che Unione Democratica per i consumatori all'interno del Gruppo Misto è l'unica componente che ha ultimato il tempo. Ringrazio i tanti amici e colleghi e i Capigruppo dei Gruppi del centro-sinistra per la grande disponibilità che non è arrivata. Ringrazio invece, senza ironia, il Gruppo di Forza Italia che mi ha messo a disposizione parte del suo tempo. La democrazia è un esercizio difficile da mettere in pratica, perché non bisogna soltanto declamarlo appropriandosi di certe attribuzioni, ma bisogna essere capaci di praticarlo, a volte in silenzio, ed io ho l'obbligo di specificare che il silenzio in alcuni casi va Presidente, con questo emendamento sottopongo al Senato una serie di questioni significative. Mi rivolgo a tutti i colleghi della Commissione giustizia,

Quando abbiamo iniziato l'esame della finanziaria in Commissione giustizia su un punto siamo stati tutti d'accordo, maggioranza

l'emendamento da me presentato ed in Aula ha invitato i colleghi della Commissione giustizia a fare memoria di un percorso condiviso; alla fine il Senato, dopo una discussione ampia e attenta, ha cancellato quella norma. Vi sembra mai possibile che, dopo un percorso democratico e partecipato iniziato in Commissione e che ha visto tutte le componenti della Commissione giustizia, e poi tutte le componenti dell'Aula, interessate ad un accordo unanime volto a stabilire che una norma come quella non può avere diritto di cittadinanza, adesso, con un decreto "marchetta" come questo, venga di nuovo cancellata quella volontà espressa in maniera consapevole dal Senato con una discussione vera? pertanto ritenuto di dover presentare un emendamento soppressivo di una norma che suona come un cazzotto negli occhi che il Governo dà al Parlamento, nel momento in cui non recepisce un'indicazione ed una volontà precisa. Il Governo crede davvero che con i decreti‑legge può tentare di turlupinare la legittima volontà espressa dalle Aule parlamentari? È mai possibile non prendere atto di quanto

gestire annullando i risultati di un confronto democratico come quello che si è svolto. Colleghi, vi chiedo di votare questo emendamento che di nuovo sopprime tale norma, luogo perché nel ragionamento che abbiamo svolto in Commissione ci siamo resi conto di come nel comparto pubblico non rendere possibile l'estensione del giudicato

l'ente pubblico ha interesse ad applicarla a tutti coloro che si trovano nella stessa condizione, per evitare di affrontare altri cento giudizi. Quindi, c'è un risparmio evidente. C'è poi un atteggiamento illegittimo, perché così facendo, vietandosi all'amministrazione pubblica l'estensione del giudicato, in effetti si fa in modo che qualcuno possa essere favorito, magari mettendo in condizione l'ente pubblico di non costituirsi al momento opportuno in giudizio, sapendo che quel giudicato favorevole nei confronti di qualcuno non potrà essere esteso.

a condividere le sue tesi e a modificare la mia idea. Penso però che non si tratti di dire sì o no ad un emendamento presentato dal senatore Manzione, ma di dire sì o no ad un'Aula che rivendica la sua dignità, ad un Parlamento che, pur se alla fine di un percorso, ha il dovere di ritenersi unico interprete di quel potere legislativo

Presidente, il divieto di estensione del giudicato è un principio fondamentale della nostra conoscenza e dottrina giuridica. Ovviamente, come ho detto in precedenza, sono disponibile ad accogliere ordini del giorno che volgano nel senso di invitare il Governo ad attuare questo rimedio, che è semplicemente di prevenzione nei confronti di ulteriori liti,

gli occhi impassibili di questo Governo sono emersi dati drammatici in ordine all'utilizzo di strumenti di finanza derivata, dei cosiddetti largamente e massicciamente utilizzati e proposti dalle banche, soprattutto nelle aree più ricche del Paese, senza alcun controllo da parte di chicchessia.

la loro crescente difficoltà finanziaria, non solo in ordine a Basilea 2 (che sta per arrivare), ma soprattutto in ordine alle difficoltà del nostro sistema delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, rispetto a un sistema del credito

verso le esigenze reali dei nostri cittadini e territori, lo copriamo colpevolmente quando talune talune banche del sistema italiano e moltissime del sistema internazionale utilizzano i nostri territori, le nostre imprese, il nostro risparmio come terreno di conquista e nient'altro. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, ma in sintesi quest'ordine del giorno prevede che il Governo superi quel limite e quella timidezza imperdonabile che si è dato in occasione dell'ultima finanziaria e affronti davvero, nonostante l'inizio di un percorso più trasparente che comunque il Governo in questa finanziaria ha reso possibile, il tema della gestione dei contratti inerenti strumenti finanziari strutturati, cosiddetti derivati, che hanno messo in ginocchio molte imprese e sotto giudizio i bilanci di molti enti locali. Invitiamo il Governo ad affrontare questo tema con tempestività. Approfitto della presenza del sottosegretario Lettieri, che ne è stato un buon testimone, per ricordare l'iniziativa e l'ampio dibattito che si è svolto in questo ramo del Parlamento durante i lavori della finanziaria,

Chiediamo qualcosa di più e ci auguriamo che anche questo tema nella presente campagna elettorale possa davvero aiutarci a trovare le utili condivisioni

non possiamo dimenticarci che non possiamo essere, questa volta con i risparmiatori ma anche con le banche: noi dobbiamo essere o a fianco dei risparmiatori o con le banche. E io invito tutti a sostenere i risparmiatori e i cittadini di questo Paese.

di nuovi. Ritengo che sia un parere finalizzato ad evitare di sottolineare l'importanza di questo emendamento. Mi rivolgo soprattutto a coloro che negli anni il Gruppo dei Verdi tra gli altri - si sono battuti per l'avvio di un programma serio di utilizzazione del bioetanolo nel nostro Paese: se non dovesse essere approvata questa proroga il programma subirebbe una battuta d'arresto difficilmente recuperabile e tutto il lavoro che è stato fatto negli anni passati a favore del comparto agricolo ma soprattutto dell'energia alternativa derivante, appunto, da sottoprodotti dell'agricoltura si vanificherebbe. È una semplice proroga dell'utilizzo di fondi già esistenti.

33, credo che il cattivo esempio della gestione dei rifiuti di Napoli sia sotto gli occhi di tutti. tratta di soldi, centinaia di milioni di euro, che non servono a risolvere il problema, ma a continuare le clientele: non ci sarà un chilo di rifiuti che andrà via dalle strade di Napoli, ma ci sarà qualche amico dei compagni che si arricchirà. Per questo chiediamo all'Aula la soppressione dell'articolo

Dovrebbe essere prorogato il termine per consentire una serie di adempimenti che sono stati introdotti recentemente che determinano anche modifiche ai *software*, da cui deriva la necessità, soprattutto per il mondo artigiano, di avere più tempo a disposizione.

questa necessità: si tratta di intervenire rispetto ad un problema che sta emergendo soprattutto per questi soggetti. Dunque, chiedo al Governo, ove non fosse possibile intervenire per via amministrativa, di intervenire per via legislativa. È vero che molte volte abbiamo dato all'Agenzia dalle entrate poteri forse superiori alla necessità, ma forse, in questo caso, sarebbe opportuno prevedere una qualche

sollecito il Governo a dare una risposta.

abbiamo varato una norma contenuta nell'articolo 2, comma 29, che sostanzialmente riduceva il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale attraverso la modifica dei parametri demografici.

e di sospendere l'efficacia della disposizione contenuta nella finanziaria. Non entro nel merito della valutazione fatta, ma pongo soltanto un problema tecnico. La dizione

il procedimento elettorale preparatorio non avviene sotto l'egida della riforma. Conseguentemente, i prefetti sono obbligati a convocare i comizi elettorali circoscrizionali utilizzando la vecchia normativa, proprio perché la definizione utilizzata è impropria. Questo emendamento serve a correggere - e non entro nel merito della disposizione - un'anomalia che creerà non pochi problemi. Infatti, la modifica introdotta dalla Camera, a parte la questione di merito, è tecnicamente scorretta. Ecco perché dico al Governo

il senatore Manzione ed altri senatori che hanno presentato emendamenti a trasformarli in ordini del giorno proprio perché la valutazione del Governo in ordine a questi aspetti, d'intesa con la Conferenza unificata, cioè con i rappresentanti delle autonomie locali, porterà sicuramente ad una migliore applicazione della norma modificata dalla Camera dei deputati.

recita: «Il Senato, visto l'articolo 49-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini, così come modificato dalla Camera dei deputati, che al fine della stabilizzazione dei precari della Croce rossa italiana le consente l'iscrizione ai registri previsti dalle leggi sul volontariato, sull'associazionismo di promozione sociale, sulla donazione del sangue e sull'immigrazione, equiparando la Croce rossa italiana che, unico caso al mondo, è nel nostro Paese ente di diritto pubblico, al volontariato e all'associazionismo, nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato e quello espresso dalla Commissione sanità del Senato in occasione dell'esame del provvedimento, considerata questa equiparazione, seppur provvisoria, sbagliata e lesiva delle attività e delle prerogative del mondo associativo italiano ed in palese contraddizione con lo svilupparsi normativo e gli indirizzi di Governo degli ultimi decenni, rappresentando inoltre un pericoloso precedente, preso atto della grande preoccupazione e della ferma protesta manifestata da tutto il volontariato e l'associazionismo del nostro Paese, invita il Governo a risolvere la vicenda dei precari della Croce rossa italiana attraverso misure diverse e più consone, evitando lo scardinamento di tutta la normativa sul *no profit* consolidata

va nella direzione di riconoscere le associazioni di volontariato soprattutto nell'ambito dei comitati locali. È questo il significato: se non partecipano al registro del volontariato, i servizi locali non possono essere riconosciuti, quindi ne restano esclusi. È questo l'aspetto che vogliamo sottolineare

di aver accettato una norma alla Camera, disconosciuta poi attraverso un ordine del giorno accolto al Senato. Questa è la gravità dell'atto che si sta compiendo in questo momento.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 21 gennaio 2008, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida: per la Regione Piemonte: Turigliatto Franco. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

proprio perché secondo me ciò è emblematico di un qualcosa che è stato consumato all'interno dell'Aula della Giunta, ma che in qualche modo dovrebbe interessare complessivamente tutta l'Assemblea. Il problema non è quello Il problema non è quello di verificare il percorso utilizzato per la Regione Piemonte, che diventa simbolo. Il problema è verificare come l'istituto dell'autodichia venga utilizzato in questo caso specifico e poi, riverberando effetti sulle altre Regioni, complessivamente in tutta la materia delle convalide. Perché? Come lei sa, signor Presidente - d'altra parte si ragionava della legge che porta il suo nome, la cosiddetta legge Calderoli c'era il problema della valutazione della possibilità di attribuire seggi a quelle liste che avessero riportato meno del 3 per cento in Regioni dove non fosse stata raggiunta la soglia del 55 Su questa problematica, che è stata la prima e che ha contraddistinto la valutazione in Regione Piemonte, c'è stato un comitato inquirente, con un'attività istruttoria molto approfondita; la Giunta, in qualche modo, è riuscita ad avere l'avallo di una serie di pareri che sono serviti a determinare una linea guida. Il problema qual è? Il problema, signor Presidente, è che, proprio per cercare di essere obiettivi (io ero il relatore per la Regione Piemonte) e al di là del fatto che nella fattispecie si ragionava dell'ipotesi che toccava il collega Turigliatto (ma questo fatto è occasionale, perché qualunque altro collega poteva essere interessato dalla vicenda), la Giunta e il relatore si sono posti il problema della possibilità di intervenire su una normativa che, quantomeno, si prestava a dubbi interpretativi che lasciavano prefigurare una prevedibile prevedibile illegittimità costituzionale della norma, proprio nella misura in cui la normativa non prevedeva una soglia specifica né in basso (in una fattispecie, infatti, il 3 per cento non veniva menzionato) né in alto nell'attribuzione dei seggi. Presidente, è diventata più attuale dopo la pronuncia della Corte costituzionale in merito alla dichiarazione di ammissibilità delle consultazioni referendarie. ammissibilità delle consultazioni referendarie. La Corte costituzionale, nel dichiarare ammissibile il *referendum* che era stato proposto, ha espressamente detto in un inciso che ci sono forti dubbi (anche se questo riguardava il merito e non l'oggetto specifico dell'ammissibilità della proposta referendaria) proprio per il fatto che non è stata prevista una soglia come tetto per l'attribuzione dei seggi e quindi per fare in modo che scattasse il premio di maggioranza.

che è rintracciabile direttamente sul sito della Giunta, proprio perché, come le dicevo in apertura, c'è stato l'apporto di tantissimi professori, cattedratici e studiosi della scienza elettorale, che hanno contribuito a darci uno spaccato. Qual è lo spaccato?

ed è stato poi corroborato da quello che la Corte costituzionale ha detto. Su questo punto, secondo me, sarebbe stato opportuno aprire una riflessione. Vedo tanti colleghi, ad esempio i senatori Boccia e Pastore, che con me si sono appassionati della vicenda. Se questo non sarà, perché consideriamo l'Aula il terminale asettico di decisioni che poi alla fine, nella situazione in cui siamo, non interessano più nessuno, quantomeno avrò lasciato agli atti, per coloro i quali dovessero cercare di comprendere qual è l'attività che è stata svolta, un riferimento che, se poi proteso verso il lavoro della Giunta, vedrà la possibilità di un approfondimento che in questa materia effettivamente c'è stato.

Con ricorso del 2 luglio 2007, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze con riferimento al provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 con cui - stabilita, nell'ambito del procedimento penale a carico del senatore Altero Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali - veniva disposta, in forza dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente senza l'autorizzazione della Camera dei deputati, nonché nei confronti del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione al provvedimento in data 4 dicembre 2006. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 8 del 14 gennaio 2008, depositata in cancelleria il successivo 18 gennaio e notificata anche al Senato l'11 febbraio 2008, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alla questione di principio da trattare. Nella seduta del 26 febbraio 2008 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, nel senso che il Senato debba intervenire in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nel conflitto citato.

Con ricorso dell'8 maggio 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto dì attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 48695/04 RGNR - n. 2764/0 6 GIP pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*ter*, n. 2) . Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 37 dell'11 febbraio 2008, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale nessun senatore intende intervenire, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. **Sono

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006. Art. 2. **Approvato**

DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006

alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007

per l'anno 2006, dando la possibilità, a chi è già decaduto, di ripresentare la domanda. L'anomalia, Presidente, non è soltanto nella violazione di un principio secco come quello della decadenza, e quindi nel fatto che venga varata una norma fotografia

facciamo i parlamentari da un po' di tempo: le risorse del 2006 come rimborsi elettorali sono già state elargite. O il provvedimento prevedeva un'ipotesi di un'ipotesi di restituzione da parte di coloro che avevano già incamerato le risorse, oppure dire che un Gruppo che non ha presentato la domanda tempestivamente viene riammesso per il 2006, tornando indietro di tre anni, significa creare il presupposto per poi per poi elargire altri stanziamenti che determinano chiaramente la violazione di una norma già di per sé illegittima. Ecco perché hanno ragione quelli che definiscono questo consesso una casta, che, tutto sommato, riesce ad attingere dalle risorse pubbliche per autoalimentarsi in maniera illegittima. Questo il senso dell'emendamento che volevo rappresentare. Questo il senso di un voto che volevo chiedere, proprio perché non mi riconosco in questo stereotipo e mi dispiace che il Governo e la mia maggioranza abbiano avallato simili scelte. Capisco che ci sono dinamiche elettorali irrefrenabili, ma capisco che non sempre c'è la disponibilità di un patrimonio (che in questo caso non è nostro personale, bensì collettivo). Atteggiamenti di questo tipo legittimano le risposte le risposte e le reprimende che vengono da giornalisti come Gian Antonio Stella. Purtroppo stiamo dimostrando di essere peggio di quella casta che è stata descritta. Ecco perché, signor Presidente, le chiedo di sottoporre a votazione il mio emendamento soppressivo dell'articolo 51-*bis*.

Grazie